il Senato non è in numero legale

nel salutare il ministro Bonino,

sul ruolo che il Ministro stesso svolge in queste ore, se ricopre o meno la sua funzione, se dobbiamo considerarlo in carica,

anche di molte delle sue idee - che noi spesso abbiamo condiviso ed apprezzato - su temi strategici del governo del Paese. Paese. Ciò che è successo ieri non può passare inosservato e noi, senza voler minimamente mancare di rispetto al Ministro, ci poniamo delle domande che ci permettiamo di rivolgere al Ministro stesso. Ieri abbiamo appreso da una conferenza stampa, resa dal partito dei Radicali, che il ministro Bonino ha rimesso il mandato nelle mani del Presidente del Consiglio, lamentando...

scelte incompatibili con la linea politica di rigore che ci viene indicata dall'Europa, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente della Corte dei conti e che vanno in controtendenza alla politica di libero mercato in cui il partito dei Radicali ha sempre creduto. Del resto non ci abbiamo trovato nulla di strano, perché abbiamo sempre

Adesso esplode irreversibilmente, secondo noi, questo contrasto e con coraggio ieri il partito radicale, ed il ministro Bonino ha posto seriamente al centro del dibattito politico la non condivisione di alcune scelte che il Governo intende attuare di qui a pochi giorni. Vi è stata la risposta del Presidente del Consiglio, che ha riconosciuto la fiducia al ministro Bonino, ma non credo si trattasse di fiducia o non, perché non mi risulta che in passato vi fossero stati dubbi o perplessità da parte del Presidente del Consiglio nei confronti del Ministro. Il tema rimane ed è ancora squisitamente politico. politico. Noi ci accingiamo a lavorare sulla legge comunitaria, con il Governo rappresentato dal Ministro. Vorremmo allora chiedere al Ministro qual è lo stato dell'arte, se dobbiamo considerarlo un Ministro dimissionario o in carica. Noi ci auguriamo di poter lavorare serenamente e tranquillamente come abbiamo fatto l'anno scorso con il ministro Bonino, persona che stimiamo e rispettiamo, però è necessario un minimo di chiarezza politica in Aula sullo stato della vicenda,

ciò che ha chiesto il collega Schifani è ragionevole. Vorremmo pertanto sapere dal ministro Bonino qual è la questione da lei posta ieri al Presidente del Consiglio, qual è stata la risposta del Presidente del Consiglio e a quale titolo oggi è presente al dibattito. Non potremmo votare una legge riguardante l'ordinamento comunitario,

Presidente, il collega D'Onofrio ha espresso in maniera esaustiva ciò che volevo dire e che non si poteva non dire, perché siamo di fronte ad un caso abbastanza anomalo. Oltre tutto, il ministro, o onorevole Bonino - questo ce lo chiarirà lei - non è neanche senatore, quindi bisogna capire se ha titolo per restare in Aula: ce lo dica rapidamente.

il ministro Fioroni si è accorto che i calcoli contenuti nella legge di riforma della maturità erano palesemente sbagliati e, dando ragione alle critiche dell'opposizione, si è anche accorto che mancavano più di 50 milioni di euro per il finanziamento della nuova maturità. Sono quindi circa 200 milioni di euro ciò che la nuova maturità viene a costare: 45 milioni di euro soltanto per il pagamento dei commissari esterni e 6 milioni di euro per quelli interni nelle scuole paritarie. Questo palese errore è stato recepito nei giorni scorsi in una ulteriore modifica di un provvedimento che giace presso la Camera, recante «Norme urgenti in materia di istruzione». Il problema grave è che sono stati tolti ulteriori 50 milioni di euro dai fondi per le scuole.

Signor Presidente, come ricorderà, ieri, non appena avuta notizia della presa di posizione del ministro Bonino, ho chiesto in Aula che il Governo venisse a riferire sullo stato dell'arte. Mi sembra di aver capito, sempre dalle dichiarazioni apparse sulla stampa,

conosciamo da tanti anni e abbiamo grande considerazione e rispetto per lei, ma non mi sembra che con quella dichiarazione del Presidente del Consiglio si sia chiarito il problema politico all'interno della maggioranza. Non è un problema che riguarda un singolo provvedimento: il ministro Bonino solleva un problema politico forte tra riformisti e massimalisti all'interno del Governo. Ora, come hanno fatto gli altri colleghi dall'opposizione, sottolineo che è opportuno che vi sia un chiarimento quando inizieremo ad esaminare un provvedimento di competenza del ministro Bonino. Non vogliamo fare nessuna forzatura, ma ci sembra che la risposta del Presidente del Consiglio non sia esaustiva; non per noi, ma - credo - per il Ministro,

che la differenza sia tra riformisti e massimalisti. A chiunque si definisce riformista auguro di segnare di sé la storia sociale e politica di questo Paese, come fece il ministro del lavoro Brodolini, che segnò un'idea di progresso e di avanzamento. Noi parliamo, e in questo sta la minaccia delle dimissioni del Ministro, di questioni rilevanti per per la vita di milioni di persone nel nostro Paese. Ci sono stati in questi giorni scienziati della politica

proposte, ad esempio prendendo atto di una difficile condizione delle donne nel nostro Paese, perché si pensa all'aumento dell'età pensionabile invece che all'aumento del montante contributivo o ad un piano straordinario per l'occupazione.

di programmazione economico-finanziaria del Governo è previsto un aumento del tasso di produttività nell'industria e una diminuzione del costo del lavoro per unità di prodotto (con cui si misura il tasso di competitività tra un Paese e un altro)

che il ministro Bonino riuscirà a sostenere, come noi le abbiamo sostenute pur non essendone convinti fino in fondo, le mediazioni che verranno proposte. So che

di costruire una mediazione avanzata su un terreno così difficile, riguardante il destino, la vita e i tempi di vita di milioni di uomini e donne.

al presente, ma sarebbe veramente un'autolimitazione incomprensibile non affrontare la questione fondamentale oggi davanti a noi. Il nostro Paese ha realizzato una riforma delle pensioni

riforme. Signor Ministro, lei dice sempre le cose giuste e poi fa sempre le cose sbagliate; o meglio, è il Governo a fare le cose sbagliate. Mi domando se lei fa la politica europea di questo Governo.

Della sua parola nessuno si fida. Non ne ha mai detta una sbagliata, non ne ha mai fatta una giusta». Signor Ministro, lei non ha mai detto una cosa sbagliata, ma il suo Governo non ne ha mai fatta una giusta. Vuole chiarire questa contraddizione?

ministro Bonino, il mio Gruppo (Verdi-Comunisti Italiani) spera che lei resti ministro, a fare bene ciò che sta facendo bene e che noi apprezziamo. Detto questo, però, con grande sincerità voglio dirle che consideriamo sbagliato l'atto che ha compiuto, e non soltanto perché, come da tempo infinito andiamo ripetendo, noi della sinistra non radicale - come lei dice, e io mi unisco a lei;

donna sicuramente di coraggio e di lealtà, avrebbe dovuto sapere, nel momento in cui entrava nella compagine governativa, a quale programma aderiva, come tutti noi sapevamo, essendo contenute nel programma anche cose che non condividiamo del tutto, insieme ad abbiamo contribuito ad elaborare. Vede, ministro Bonino, noi non siamo d'accordo soprattutto perché sulla questione pensioni‑scalone (lo scalone è una mascalzonata sociale che ci ha lasciato il Governo Berlusconi)

parlando: di qualcosa che riguarda meno di 800.000 lavoratori che hanno cominciato a lavorare da ragazzi. È una vergogna la controinformazione che si sta facendo. Per questo, ministro Bonino, pur rispettando il lavoro che lei ha fatto nella sua vita e le lotte che ha sostenuto per i diritti civili, voglio esprimerle il mio dissenso, amichevole se vuole, ma totale, per l'atto che ha compiuto, sperando che ci ripensi.

A questo intendo attenermi sostanzialmente e formalmente, nella pienezza delle mie funzioni. A questo e non altro. Per il resto, è aperto un dibattito pubblico, limpido, e non ci sono né novità né decisioni. Quando e se ci saranno, il Governo ed io personalmente non mancheremo di rispondere alle eventuali sollecitazioni di questa o di altra Camera. Vi ringrazio.

e soltanto per la sua presenza formale. Noi possiamo passare all'ordine del giorno e andare avanti; abbiamo anche, tra l'altro, precedenti recentissimi, oltre che indicazioni chiare del Regolamento.

in questa legislatura. Molte cose che a noi erano proibite oggi sono lecite. Vorrei capire se è cambiata la Costituzione, se è cambiato il Regolamento del Senato o se, semplicemente,

soprattutto per l'Aula - è significativa del disagio politico presente all'interno della maggioranza. La sua dichiarazione,

Io sostengo che questa mattina il ministro Bonino non ha reso dichiarazioni. Con moltissima sobrietà e chiarezza, ha risposto a diverse sollecitazioni di senatori che chiedevano in che veste è qui. La sostanza è che ha detto di essere qua in veste di Ministro, non negando che c'è poi un dibattito politico. Questo è il fatto che mi spinge ad attenermi all'articolo 99. L'articolo 105 c'è e lo conosco bene. Se ci sono dichiarazioni, i lavori si svilupperanno come previsto dall'articolo 105. Voglio rassicurare che non intendo forzare alcunché. Vi ringrazio.

mi sembra che lei oggi applichi un criterio assai diverso da quello adottato in una recente qualche ora fa, qualche giorno fa, lei ha considerato come politicamente rilevanti, e quindi tali da legittimare una discussione e un voto separato in quest'Aula, emendamenti dal contenuto sostanzialmente identico. Ricordo bene? In quella occasione ci disse che il criterio adottato era quello di garantire il massimo di possibilità di espressione per l'Assemblea parlamentare arrivando in qualche caso

che non riesco a capire: o si applica un criterio estensivo o si applica un criterio riduttivo; o si applica un criterio formale o si applica un criterio di contenuto. Non si può, secondo la convenienza, applicare una volta un criterio formale e un'altra un criterio di contenuto.

«Nel contesto in cui siamo, ho ritenuto doveroso, necessario e urgente rimettere alla valutazione del Presidente del Consiglio se il mio permanere nel Governo sia ancora utile o per lo meno compatibile con le scelte che lui sia appresta a fare e a comunicarci». Cosa significa questa frase? Lei ha rimesso le deleghe oppure no? Forse è la solita questione all'italiana, e ne abbiamo viste tante, in questi giorni: l'Associazione nazionale magistrati che preannuncia uno sciopero e poi ovviamente non lo fa, questa sua dichiarazione, l'episodio di ieri che effettivamente per certi versi non è stato del tutto chiaro in quest'Aula.

il Ministro, un rappresentante del Governo, è qui a pieno titolo, a pieno effetto, con quale cogenza rilascia i propri pareri sugli emendamenti e sugli articoli, oppure se è qui tra coloro che sono sospesi. La sua dichiarazione, peraltro molto stringata, è stata anche criptica, non si è compreso nulla. Vorrei capire esattamente quali sono le peculiarità e le prerogative dell'onorevole Bonino in questo momento in quest'Aula.

non si può dire che siamo nell'ipotesi alla quale lei fa riferimento. Non si può dimenticare, infatti, che ieri il senatore Matteoli ha posto il problema delle dimissioni in diretta del ministro Bonino. Il ministro Bonino con quella dichiarazione non si è richiamata alla circostanza che si sta discutendo un provvedimento di legge e che si è chiusa la discussione generale; al contrario, ha fatto una dichiarazione eminentemente politica, ovvero ha dichiarato di trovarsi in una posizione "disimpegnata", per la quale la sua presenza, come dire, c'è e non c'è. c'è. Il ministro Bonino non giura e non dichiara la sua fedeltà nel nostro sistema politico al Presidente del Consiglio: lo fa rispetto alla Costituzione e - siamo in una democrazia parlamentare - al Parlamento. Quindi, la sua dichiarazione è impegnativa, lascia intendere che allo stato si sente "sospesa" e che ancora non ha deciso il da fare, anzi addirittura aggiunge che lo spiegherà in un'altra occasione,

dichiarato di restare in attesa. Questo è un fatto politicamente rilevante, del quale l'Aula non può non discutere. È un fatto che rileva per il rapporto che esiste in una democrazia parlamentare tra un Ministro e il Parlamento. Non si può dire ai senatori: aspettate, adesso vedremo, quando si deciderà, quando si capirà quale provvedimento sulle pensioni sarà preso, se il ministro Bonino insisterà, svolgeremo il dibattito, perché la nostra è una democrazia che si svolge giorno per giorno ed è, o dovrebbe essere, una democrazia responsabile. Per questo ritengo con forza che su questo tema si deve aprire un dibattito e che il ministro Bonino ci deve spiegare perché ha ritenuto di dimettersi e perché oggi in quest'Aula dà una risposta blanda, una risposta di attesa, cosa c'è di mezzo, cosa ci si attende. Il Parlamento ha tutto il diritto di intervenire in questa fase delicata della vita politica italiana. Non è possibile che tutti

proprio ai sensi dell'articolo citato.

comunista reazionario, che ha imparato ad essere reazionario a 17 anni, quando ha cominciato a frequentare una persona, arrivata in Sicilia al mio paese, che si chiamava Danilo Dolci, per fare i primi digiuni per sostenere una famiglia di pescatori e che cominciò poi, e coinvolse noi ragazzi, a fare lo sciopero della fame e lo sciopero alla rovescia, che consisteva nell'andare a lavorare a sistemare le trazzere malgrado non ci fossero le autorizzazioni, ma per rivendicare un lavoro. A quelli più adulti - io ancora ero minorenne - quell'operazione costò un processo che vide i i più grandi avvocati di allora e lo stesso Calamandrei venire a difendere Danilo Dolci e tutti quei banditi reazionari che avevano fatto lo sciopero alla rovescia. Sono cresciuto in quella storia, con quella scuola (l'ho fatta nella CGIL, per tanti anni): il confronto di merito sulle posizioni assunte di volta in volta nel e dal sindacato ovviamente ha dato luogo anche ad aspri scontri politici. Se dovessi ricordare - ed il presidente Marini se lo ricorderà meglio di me, perché credo l'abbia vissuto in prima persona - un tentativo d'accordo sulle pensioni, portò, attraverso una consultazione di tutti i lavoratori, i segretari confederali di allora (Lama, Storti e Vanni) a ritirare una firma, perché le loro organizzazioni non avevano dato il mandato. L'accordo sulle pensioni si fece nel 1969, due anni dopo, in seguito allo sciopero generale:

che le dichiarazioni rese stamattina in Aula, nella pienezza delle responsabilità della sua funzione e della sua carica, non determinino alcun elemento di ambiguità,

che la ministra Bonino viene qui a rappresentare il Governo sulla politica comunitaria, sto a questo; sul resto (la lotta ed il confronto politico), il dibattito è aperto, ma la strumentalizzazione certamente no.

ieri, apprese le notizie dell'ipotesi di dimissioni del ministro Bonino, abbiamo chiesto immediatamente, tramite il presidente del nostro Gruppo, senatore D'Onofrio, un chiarimento urgente al Governo. Lo abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio tramite la sua autorevole Presidenza, ma tutto ci saremmo aspettati meno che trovarci in quest'Aula, in questo costretti ad «estorcere» un consenso per poter parlare con il linguaggio della politica, con il linguaggio istituzionale. Ci saremmo aspettati, colleghi senatori, che il Presidente del Senato avesse convocato il Governo a riferire al Senato della Repubblica quello che stava accadendo. Abbiamo visto, invece, che le cose sono andate in modo diverso con un tentativo di non discutere, e se oggi, in questo momento, stiamo parlando è soltanto perché la sensibilità del Presidente, non il diritto di quest'Aula di discutere, ci concede la possibilità di interloquire sui problemi del nostro Paese.

del nostro Paese, come mai ci siamo trovati in questo dibattito e se concorda con noi che il Governo risponde al Parlamento e il Parlamento risponde al popolo, perché questa è la prima regola con la quale dobbiamo in qualche modo convivere e la nostra posizione politica deve marcare questo senso di responsabilità. Nella democrazia parlamentare ci sono delle regole: lei ha dato inizio ad un dibattito e non vorremmo che tale dibattito, dopo essere stato oggetto di una iniziativa dei giornali e delle agenzie di stampa, fosse sottratto alla discussione dell'organo sovrano che è il Parlamento italiano e quindi il Senato della Repubblica. Lei ci ha detto in questa che non c'è nessuna novità e nessuna decisione, mentre noi sappiamo che ci sono state lettere: l'attività del Governo e di un suo Ministro non sono cose riservate ad una maggioranza. Io credo che lei abbia il dovere di dire all'Aula ciò che ha riferito al Presidente del Consiglio, a meno che non siano cose private, non siano, cioè, cose che riguardano la sfera privata dei rapporti tra lei e il Presidente del Consiglio. Abbiamo anche ascoltato le considerazioni del senatore Bonadonna senatore Bonadonna e di altri colleghi che sono intervenuti, dei comunisti che in quest'Aula si sono richiamati anche all'orgoglio delle attività reazionarie, come ricordava, appunto, il collega Bonadonna al quale

persone che hanno sulla politica estera, sulla politica comunitaria, sulla questione delle pensioni - come l'onorevole Bonino ha manifestato da sempre - diversità di vedute, anche nello stesso Governo, non abbiano la forza politica di mettere l'interesse generale prima dell'interesse di una coalizione, di una maggioranza. Questo è il nodo, e se è vero che l'antipolitica, in questo momento, prevale nel nostro Paese, noi dobbiamo rafforzare, con onestà politica e intellettuale, le ragioni della politica stessa, prima di tutto rispettando il Parlamento, rispettando le istituzioni, rispettando i Regolamenti, rispettando cioè quel momento politico particolare che rappresenta il popolo italiano. italiano. Con questo sentimento, signor Ministro, invito lei e il Presidente del Consiglio a chiarire al Parlamento italiano, e quindi ai cittadini italiani, qual è la condizione reale. Noi siamo preoccupati perché non sappiamo se c'è ancora una politica europea nel nostro Paese,

e concludo, signor Presidente - se c'è ancora la forza e la capacità, da parte di questa maggioranza, di questo Governo, di poter dare al nostro Paese un minimo di risposta politica sui temi che riguardano gli interessi generali. Mi sembra che questo non ci sia. Mi sembra che l'ultimo atto del ministro Bonino sia in linea con l'incapacità di dialogare anche nelle istituzioni, con tutto il rispetto per il Ministro, alla quale riconosciamo riconosciamo quella intuizione politica di capire che con questa maggioranza non si va da nessuna parte, però prima di questo c'è il rispetto delle istituzioni. Signor Presidente, il Regolamento lo sappiamo leggere tutti;

parlare se dobbiamo approvare o respingere emendamenti che il Governo sarà costretto comunque a ritirare se non vorrà fare la figuraccia di porli ai voti e quindi di vederli bocciati.

signori del Governo, colleghi senatori, mi sarei aspettato, dopo le dichiarazioni del Ministro di ieri pomeriggio, il bombardamento delle televisioni e della stampa di questa mattina, che il dibattito non si svolgesse oggi in quest'Aula.

ed eventualmente ci sarà comunicato quello che succederà. Non funziona così. Un rappresentante del Governo rappresenta sempre l'Esecutivo in quest'Aula, indipendentemente dalla singola questione che viene a trattare. Il Governo è un organismo collegiale e i Ministri che sono seduti al banco del Governo lo rappresentano in qualunque momento del dibattito. Se adesso succedesse all'esterno qualcosa che non

Le parlo avendo apprezzato nella storia della mia vita le posizioni che lei, il suo partito e il suo movimento hanno rappresentato. Le dico di più; quando in numerose occasioni ci avete detto: o ci scegli o ci sciogli, io sono tra quelli che vi hanno scelto,

rappresentare una coalizione al Governo è un altro esercizio, che si compie nella collegialità espressa dal Consiglio dei ministri che manda ogni singolo Ministro in Parlamento. La invito ancora una volta, se fosse possibile, a chiedere lei al Senato di rimandare questa discussione, a mettersi nella condizione di avere nel Consiglio dei ministri il chiarimento che lei ha chiesto e ancora non ha avuto dal Presidente del Consiglio. In seguito, quando avesse trovato l'accordo all'interno del Consiglio dei ministri, la invito a presentarsi nella sua pienezza di rappresentanza al Parlamento per dibattere un argomento così delicato. Quello che stiamo facendo oggi è un esercizio che diventa un tecnicismo che niente ha a che vedere con la politica e con le regole della politica con la "P" maiuscola, che regolano la vita dei Governi e il funzionamento dei Parlamenti.

prima di intervenire sulla legge comunitaria e sulla relazione circa la partecipazione italiana all'Unione Europea, mi prendo la libertà di esprimere a titolo personale, ma credo con un giudizio che non è soltanto individuale, il sincero appezzamento

Non vado oltre, signor Presidente, per rispetto alle sue direttive. Se fossi indisciplinato cadrei nella tentazione Senatore, non sia indisciplinato questa mattina. ZANONE *(Ulivo)*. ...di comprendere la serietà - mi lasci dire soltanto questo - dell'allarme o del preallarme espresso ieri dal ministro Bonino. Lei però mi vieta di andare oltre e, siccome siamo nell'anno delle celebrazioni garibaldine, io obbedisco, anche perché non mancheranno ulteriori occasioni di occuparci di questo problema.

in vista della Dichiarazione di Berlino, che fu il primo e non trionfale momento pubblico del semestre tedesco.

insieme ai senatori dell'intergruppo federalista, si provvide a presentare un'altra proposta di risoluzione, il 20 giugno, nella speranza che fosse possibile, come nel primo caso, arrivare ad una presa di posizione del Senato che esprimesse al Governo le aspettative dell'Assemblea nei confronti di quei decisivi appuntamenti con il processo di costruzione dell'unione politica.

l'idea dell'Europa come cittadinanza comune e l'idea dell'Europa come negoziato delle convenienze particolari. Si è svolta cioè una discussione fra coloro che intendono l'Europa come una cittadinanza comune e coloro che intendono l'Europa come un luogo per negoziare le proprie particolari convenienze.

La Presidenza tedesca, sulla quale si affidavano grandi aspettative da parte di tutto il mondo europeista, ha svolto il suo mandato semestrale forse senza eccezionali capacità inventive e creative, ma con una precisione teutonica, riuscendo quindi ad ottenere un mandato negoziale che ha il merito, se vogliamo dirlo, di essere formulato in termini precisi e delimitati. Questo dà qualche ragione di limitato ottimismo circa la Conferenza intergovernativa che si deve concludere entro l'anno, perché lascia sperare che la conduzione del semestre portoghese, che deve portare a concludere i Conferenza entro ottobre, non riapra le questioni che a Bruxelles sono state trattate e decise in forme semplificate e che si possono anche comprendere, data l'esigenza politica da parte di molti Stati dell'Unione di evitare il pericoloso il pericoloso ricorso a nuovi *referendum* nazionali. Tutto questo però ha un prezzo, ed è un prezzo gravoso per l'idea dell'Europa come cittadinanza, perché il risultato che è stato raggiunto in questo modo non riavvicina l'Europa ai cittadini. Mi limito a citare quattro o cinque voci della lista dei prezzi che sono stati pagati per arrivare al mandato negoziale, al superamento della situazione di stallo, che era ormai arrivata ad un punto cronico, e al riavvio verso il nuovo Trattato, che non sarà più il Trattato della Costituzione, ma sarà il Trattato della riforma. Il primo prezzo è il rifiuto dei simboli: nessun riconoscimento costituzionalizzato per il motto, per la bandiera, per il nome di legge dei provvedimenti europei, per l'inno. l'inno. È piuttosto spiacevole che si sia negato un riconoscimento costituzionale anche all'inno di Schiller, che noi chiamiamo "Inno alla gioia", ma che, se non ricordo male, in origine si chiamava "Inno alla libertà". Ebbene, si dice che tutto questo è soltanto un fatto formale, simbolico, che non ha un costo sostanziale perché tutte queste consuetudini, questi simboli dell'Europa resteranno nell'uso. Però, io non sono di questo avviso, solo ove si consideri il significato della parola: "simbolo" significa ciò che mette insieme, è cioè il segno dell'unione. ciò che lascia molto delusi gli europeisti è il fatto che si siano negati i simboli per negare l'unione! Questo è il primo prezzo pagato dalle conclusioni di Bruxelles! che si è abbandonato il Trattato costituzionale dopo anni di lavoro e di negoziati. Noi tutti ricordiamo la grande opera, l'intelligenza e anche la pazienza che per l'Italia Giuliano Amato ha dedicato ai lavori della Convenzione. I risultati della Convenzione erano un compromesso; si arrivò poi ad accettarli da parte dei Governi con un altro compromesso, quindi con una graduale e scalare riduzione delle delle prime prospettive alquanto vagamente federalistiche; però vi era un Trattato costituzionale, pur se pletorico, inutilmente complicato e numeroso nella sua articolazione; tuttavia è stato abbandonato. Anche in caso, si è abbandonato il Trattato costituzionale ma, in realtà, per abbandonare l'idea di una Costituzione. Questo sarà grave perché aggraverà lo squilibrio tra il progressivo allargamento dell'Unione - destinata ad espandersi ancora verso il mondo balcanico, domani verso la Turchia fino all'Europa a 30, 33, 34 componenti - e la sua profondità istituzionale. Stiamo pagando in termini di ampiezza quello che non riusciamo ad acquisire in termini di profondità. terzo prezzo pagato è l'arretramento del principio della libera concorrenza non falsata: questo era nel Trattato ed è stato relegato in una protocollo aggiuntivo. E mi ha abbastanza sorpreso che il fatto sia stato commentato con una certa accettazione realistica da parte di Mario Monti, il commissario che più si è adoperato proprio nell'esercizio del governo della concorrenza nell'ambito della Commissione europea. Non credo che anche questo sia un prezzo lieve, perché il principio della concorrenza non falsata è una delle radici della costruzione europea, che già compariva nei Trattati di Roma di cinquant'anni fa.

per celebrare l'esordio, in campo europeo, del presidente francese Sarkozy. Altro prezzo: l'inclusione, solo per richiamo, della Carta dei diritti. Anche questo è un punto importante, perché nella Carta dei diritti si vedeva, forse con un eccesso di illuminismo, il tentativo di estendere l'adozione dei diritti civili e sociali e di cittadinanza al di là degli Stati-Nazione, cioè in una dimensione effetti costituzionalmente sovranazionale. La Carta dei diritti acquisirà l'efficacia giuridica che nel Vertice di Nizza non gli era stata

e celebrare l'esordio del presidente francese Sarkozy, a questa riduzione dei margini della Carta dei diritti si è ricorso invece per celebrare l'esodo del *premier* inglese Blair.

rinvio in un arco ragionevole di una decina di anni, stabilito per accontentare i capricci del Governo polacco,

si è scelta la strada dell'Europa della cittadinanza comune ma l'Europa delle convenienze nazionali. A fronte di ciò, bisogna pur dire che gli obiettivi istituzionali che avevamo segnalato nel nostro progetto di risoluzione del 20 giugno, alla vigilia del Vertice di Bruxelles, sono stati, almeno in parte, conseguiti e non si può minimamente sottovalutare il rilievo dei risultati ottenuti in materia di supremazia del diritto comunitario sulle legislazioni nazionali, di riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione, di abbandono del sistema dei pilastri, di assegnazione della vincolatività giuridica alla Carta dei diritti (di cui ho detto), di elezione di un Presidente del Consiglio stabile (in luogo dell'attuale turnazione semestrale), di nomina di quello che non sarà un Ministro degli esteri ma comunque un Alto rappresentante degli affari esteri e della politica di sicurezza, dotato di un proprio servizio relazioni esterne, e, infine, di estensione del voto di maggioranza (sia pure con le ampie clausole di rinvio di cui già ho detto). Dunque, qualcosa è stato ottenuto, quanto basta per evitare che quella che è stata, in termini di prospettiva europea, una mezza sconfitta diventasse una disfatta totale.

di questa strana armata che avanza fermandosi quando si stanca la retroguardia. Tutte le avanzate dell'Europa si fermano quando la retroguardia lo decide. Questo deve dirci qualcosa sul futuro. Mi sembra si tratta di una ragione quasi obbligatoria per riconoscere e accettare che, se l'Europa vuole andare avanti un po' più alla svelta, per non restare sempre indietro rispetto ai fatti che accadono e che richiederebbero la sua presenza sulla scena internazionale e mondiale, deve

sempre naturalmente lasciando aperto uno spazio all'adesione dei ritardatari che decidano di aggiungersi al convoglio in un secondo tempo. Qual è allora il duplice nuovo obiettivo che si pone? Anzitutto, quello di sostenere la Presidenza portoghese perché i lavori della Conferenza intergovernativa si concludano entro l'anno, evitando che si riaprano ci sono già da parte della Polonia segni piuttosto preoccupanti in questo senso in merito a questioni che si vogliono riaprire per ottenere nuovi compromessi al ribasso. Occorre contrastare tale eventualità. occorre non disattivare il processo verso la costruzione dell'Unione politica che, certo, a Bruxelles ha segnato una battuta di arresto sotto il profilo della costituzionalizzazione, con un vero e proprio atto di abbandono, e che, tuttavia, deve riprendere nelle forme in cui ciò è possibile: cercando, se sarà possibile trovarlo, un nucleo di avanguardia comprendente i sei Paesi fondatori e così risolvendo

Ciò che connota la nostra Nazione in senso positivo agli occhi dell'Europa è proprio questa tradizione europeista e federalista, che fa parte della nostra migliore cultura politica e civile fin dagli anni

Napolitano. Signor Presidente, il profilo europeistico del Governo, sicuro nell'azione svolta e nella stessa titolarità dei suoi principali Ministri, ci rende fiduciosi sull'azione di anticipazione e avanguardia che il Governo italiano continuerà ad esercitare, in vista della scadenza del 2009 che sarà, nelle prospettive dell'Unione Europea, il momento della verità.

il Gruppo dell'UDC interviene in questo importante dibattito sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, sulle modalità e i termini

perché siamo convinti che l'Italia abbia dei valori fondamentali da sostenere e da portare avanti e che, in dote all'Europa, noi possiamo portare tante specificità ed eccellenze italiane.

Quando parlo di specificità e di eccellenze italiane, parlo del valore delle nostre politiche agricole e delle nostre intelligenze, del valore di superpotenza, che noi siamo in termini culturali, e del patrimonio umano, che possiamo e abbiamo certificato nel mondo, prima, durante e dopo l'ultimo millennio, in termini culturali e scientifici. Con questa consapevolezza, signor Ministro, vogliamo offrire il nostro contributo

Il senatore Zanone ha ricordato poco fa quanto in Italia è stato fatto per raggiungere il valore europeo e quanto si potrebbe ancora fare; quanto la mediazione politica - aggiungo io probabilmente non porta a casa dei grandi risultati, perché i valori a cui facevamo riferimento prima molte volte rimangono sul tavolo del negoziato politico (mi riferisco alla difesa della nostra specificità).

noi abbiamo apprezzato il fatto che nel provvedimento ci siano molti aspetti che condividiamo. Però manca, sostanzialmente, qualcosa anche dal punto di vista della *better regulation*, della semplificazione amministrativa, di tutte le questioni innovative che in Europa, anche durante il precedente Governo, io stesso, come Ministro della funzione pubblica, ho portato avanti con il provvedimento "taglia leggi"

che i pieni adempimenti europei sul "taglia leggi", per semplificare la vita dei cittadini e delle imprese europee, potevano essere un'altra via italiana, una via da seguire, ed abbiamo indicato questa specificità italiana, riconosciuta in Europa, come linea e come vocazione: quella di avvicinare il cittadino utente alla pubblica amministrazione. Ma non solo questo, signor Ministro. Abbiamo voluto indicare nella nostra proposta di risoluzione anche elementi importanti sul silenzio‑assenso su tutto quello che noi possiamo portare in dote all'Europa e, ovviamente, il tema più significativo, che sottolinea la vocazione di un Governo animato da valori, non di un Governo tecnico. Io credo che ella, signor Ministro, rappresenti un Governo animato da valori, che io condivido in parte su alcuni aspetti. Ma, probabilmente, su tutte le questioni legate ai valori della storia della nostra Europa c'è una forte carenza. Come veniva ricordato in quest'Aula, in un momento come questo, in cui il bipolarismo muscolare impedisce all'interesse generale di prevalere, cui il bipolarismo in questo momento storico è diventato da elettorale anche "bileaderistico", noi abbiamo delle difficoltà a rappresentare tutti i problemi del ceto medio europeo, di quella comunità europea che nella stragrande maggioranza vuole essere governata con il buonsenso e con l'arte della politica e che vuole rimettere le estreme (quindi le specificità estreme, gli estremismi di destra e di sinistra) nel loro posto naturale, cioè all'opposizione. Allora, queste vocazioni, i valori e l'ispirazione cristiana dell'Europa non sono un riconoscimento per il futuro: il riconoscimento della nostra storia, soprattutto perché con i valori cristiani e i valori laici si può immaginare un futuro governo europeo e degli Stati che lo compongono. Quello che ci preoccupa è il laicismo ideologico, che prevale in questi documenti, perché omettere la nostra vocazione, la nostra storia significa portare l'acqua a quel laicismo ideologico che diventa un neopaganesimo europeo. Su questo dobbiamo tracciare le differenze. Non è il colore delle nostre casacche che ci divide, colleghi senatori, ma sono le differenze sul modello di vita europeo, sui valori, sul futuro delle nuove generazioni;

come i nostri figli e chi verrà dopo di noi dovranno vivere, con quale modello di vita, con quali valori, con quale Europa. L'Italia gioca un ruolo importante. Il primo ruolo non può essere quello di giocare la grande politica europea nascondendo le proprie vocazioni, la propria storia, come se avessimo vergogna di riconoscere che il nostro Paese può dire molto nel valore dei valori che rappresenta.

le politiche di attuazione del Consiglio ECOFIN, su tutto quello che dobbiamo fare; sulla sensibilità che lei ha posto anche in questi giorni all'attenzione del Governo presieduto dall'onorevole Prodi, sulla questione della riforma pensionistica, per garantire la sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici, anche nell'interesse delle giovani generazioni. Non dobbiamo infatti dimenticare che noi non abbiamo ereditato questo mondo, questa Europa, ma l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli e dobbiamo riconsegnarla loro con grande attenzione e senso di responsabilità.

non è un appoggio ideologico, ma fondato sui fatti concreti. Se deve differenziarsi in questo Parlamento dall'estrema sinistra, dalla sinistra radicale, che vuole ovviamente portare a casa risultati diversi dall'interesse generale della nostra Comunità europea, lei può farlo perché ha il sostegno di quell'ampia fascia culturale e politica che in questo Parlamento prevale, ma che ha bisogno di avere delle risposte. Le risposte non possono essere effimere, ma devono essere nell'interesse supremo del Paese.

Signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, care colleghe, c'è un interrogativo che non posso nascondere travolge in questo momento, in cui stiamo per confermare la nostra adesione ai princìpi comunitari, insomma all'Europa: a quale Europa noi oggi confermeremo di appartenere? All'Europa dell'enfasi con cui abbiamo celebrato in quest'Aula il cinquantenario del Trattato di Roma o all'Europa - o alle macerie di Europa - scaturita dall'ultimo Consiglio di Bruxelles? Non voglio essere catastrofista, ma appare chiaro a tutti, come detto dal collega Zanone poco fa, che per chi sperava che dall'ultimo Consiglio del semestre tedesco scaturisse

di processo di integrazione sociale, di normative da armonizzare, di mercato interno, di concorrenza, di politiche comuni, ma soprattutto di coesione economica (ancora una volta economica). Ma quale coesione può farsi strada nel popolo europeo (che non esiste, è un insieme di popoli) se non interviene anche quella che stavamo per ottenere, ossia la coesione politica che la Costituzione ci garantiva? Il collega Zanone, pur nella severità della sua analisi, a volte impietosa, ha detto che abbiamo osservato una battuta d'arresto sul percorso verso il federalismo, verso un'Europa veramente unita e coesa. Ma io sono ancora più drastico. La storia non solo si è fermata, ma ha fatto un passo indietro, un grave passo indietro, soprattutto se andiamo a recuperare non solo l'enfasi delle celebrazioni in quest'Aula di poche settimane fa, ma anche l'entusiasmo con cui nella primavera del 2004, in Campidoglio, non lontano di qui, fu firmata quella che allora nessuno si vergognava di chiamare Carta costituzionale costituzionale da tutti i 27 Paesi che oggi compongono l'Unione Europea. Alcuni Paesi erano ancora in veste di candidati, ma nessuno si tirò indietro e il tutto accadde, avvenne - lo ricorderete - in una cornice di entusiasmo, di bandiere azzurre, di stelline dorate, di inni alla gioia sprecati in ogni cerimoniale, cose che da quel giorno sono state messe nel retrobottega e che il Consiglio europeo di Bruxelles ha cancellato. Ora, come si fa a parlare (lo ha fatto anche Angela Merkel), di un risultato positivo o - peggio - di un successo del Consiglio europeo di Bruxelles, per il solo fatto che si è riusciti ad evitare la diaspora dei polacchi o l'uscita di altri Paesi di recente costituzione come Paesi comunitari? Mi chiedo: vale di più ciò che si è perso di quello che c'era prima di questo Consiglio o vale di più ciò che si è recuperato, che si è conservato, che è veramente il minimo rispetto a quello che preesisteva? E allora non so come si faccia a parlare di successo solo perché si è ottenuta la convocazione di una Conferenza intergovernativa, che non potrà fare altro che mettere in ordine le macerie di una carta costituzionale ormai relegata al ruolo di semplice documento riformatore di Trattati. Questo è il grave passo indietro. Avevamo concordato una Carta costituzionale, ma il primo punto approvato da quel disastroso Consiglio dei ministri è che mai più in Europa si potrà chiamare Costituzione o costituzionale qualsiasi documento comunitario. L'occasione di avere una Costituzione si è trasformata, è stata ridimensionata in una delle molte previsioni di cui il Trattato è stato fatto oggetto in questi ultimi Ma non è il solo passo indietro che è stato compiuto, altri colleghi ne hanno ricordati diversi. A me preme soprattutto evidenziare un tono generale di rinuncia alla costruzione, al consolidamento di di un clima, di una politica comunitaria anche per l'appartenenza dei nuovi Paesi, che hanno profondamente deluso. Hanno fatto notevoli insistenze prima della loro adesione per poter avere l'*acquis communautaire* e un volta all'interno hanno gettato la maschera ed hanno manifestato tutta la loro immaturità a partecipare ad un sodalizio come quello dell'Unione europea. Dove sono finiti lo spirito e la capacità costruttiva dei membri della convenzione che tra il 2002 e il 2003, in 18 mesi di lavoro entusiasmante, riuscirono a concordare un difficile testo di Carta costituzionale? Eppure erano persone di grande statura politica, morale, giuridica, i rappresentanti di tutti i Paesi e di tutti i Parlamenti, oltre che del Parlamento europeo. Ma possibile che quelle 105 persone che avevamo delegato come rappresentanti, i migliori della nostra Europa, abbiano sbagliato tutto, ma non solo perché non sono riusciti a concordare le radici cristiane, il preambolo e così via, ma anche tutto il resto del loro lavoro è stato miseramente buttato alle ortiche? Questo perché sono prevalsi, come sempre, i Paesi tradizionalmente euroscettici, come sono stati sempre definiti, ma con l'aiuto di Paesi di nuovo scetticismo che viene dall'Est. Hanno vinto gli inglesi, ha vinto Tony Blair; infatti, il rifiuto della carta dei diritti fondamentali non era nuovo da parte degli inglesi, ma riuscire a togliere l'intera parte seconda della Costituzione, a relegarla a semplice riferimento di qualsiasi cultura o documento è una botta, è una sconfitta per tutti coloro che da Nizza avevano creduto veramente in una svolta di ideali europeistici: ideali di mercato ad ideali di comunità sociale, di valori umani e di valori condivisi. Tutto quello è stato considerato superfluo, superato, o peggio, inutile. Poi, ancora, il tanto auspicato Ministro degli esteri europeo, da inviare in tutto il mondo nei focolai di conflitto con una patente finalmente vera, credibile, di rappresentatività autorevole, di un qualcosa di coeso, di convinto di poter esercitare un proprio ruolo anche a livello internazionale, questa figura è stata abbattuta; peggio ancora, ne avevamo due, Solana come alto rappresentante e la Walder Ferrero come commissaria per le politiche estere, mentre ora ci sarà un solo personaggio a rappresentare quello che rimane della politica estera europea, una sorta di ambasciatore senza credenziali. Ha vinto Tony Blair, ha vinto la politica di coloro che intendono conservare egoisticamente ai Governi nazionali qualsiasi intervento di politica estera, che è il peggio di tutto: parlare con 27 voci diverse sullo scenario mondiale. Poi, ancora, come ha accennato qualche oratore precedente, il voto a doppia maggioranza, che darebbe maggiore credibilità alla democrazia in Consiglio scatterà solo, se va bene, nel 2017. Fino ad allora l'egoismo nazionale continuerà a prevalere sullo spirito comunitario: ma i polacchi, che hanno 40 milioni di cittadini e pretendono di contare quanto la Germania che ne ha il doppio, dov'è in questo atteggiamento un minimo spirito comunitario, una capacità di dialogo, di capire che, se si vuole far parte di una famiglia, occorre abbandonare o rinunciare ad una porzione del proprio egoismo per condividere le posizioni di tutti gli altri? Infine, una questione non secondaria. Diciamo la verità, l'inno alla gioia l'avevamo imparato tutti, lo potremmo perfino cantare se ci impegnasse un pochino. Non lo potremo più fare, se non il 9 maggio in occasione della festa dell'Europa, o in qualche circostanza di colore, ma guai se qualcuno dovesse mai immaginare che questa musica, ormai entrata nel sangue e nella fantasia degli europei, dovesse mai assomigliare ad un inno nazionale, non è possibile. E così, la bandiera alla quale siamo ormai abituati, c'è un'invasione di stelline e di bandiere azzurre ovunque, è semplicemente un oggetto decorativo ma non simbolico, perché chiaramente non potrà rappresentare più nulla di quello che sognavamo noi romantici costruttori della Costituzione. Accanto a questi sei o sette motivi di pessimismo, uno soverchia tutti: l'*opting out*, una formula terribile attraverso la quale ogni Governo potrà da adesso in poi prendere dall'Europa ciò che gli conviene e potrà rinunciare, rifiutare tutto quello che implica un impegno, qualcosa di oneroso o di fastidioso. Sarà la classica Europa *à la carte* che tutti credevamo di aver ormai abbandonato o relegato ai tempi della costruzione del cantiere dell'Europa. non solo l'edificio è stato abbattuto, ma sono stati allontanati anche tutti i possibili interventi per realizzare un nuovo cantiere. Due cose soltanto

del minimo certamente): l'abolizione dell'assurda Presidenza semestrale per incaricare finalmente per due anni e mezzo un autorevole Presidente del Consiglio, che dia continuità

Una bella utopia riuscire a ridurre a 15 i commissari, se le premesse sono quelle che abbiamo visto a Berlino. Vorrei

fuori sempre 9: se dovesse toccare ai polacchi, ai cechi, a qualche Paese di fresca acquisizione, o agli italiani, non vorrei essere in quel momento al centro del dibattito. Infine, vorrei chiudere il mio intervento richiamando proprio la parte conclusiva della relazione del nostro relatore, una frase che, dopo tanto pessimismo - mi scuso con chi non è così accorato sui temi minimo di speranza. Le ultime parole della relazione del senatore Manzella sono le seguenti: «Nel difficile momento che attraversa L'Unione europea, l'Italia è chiamata ancora una volta a svolgere, oggi più che mai, la sua storica funzione di "Paese federatore". Un Paese che -sia pur conscio delle sue debolezze strutturali e interessato a superarle, specie per quanto riguarda il risanamento dei conti pubblici - abbia però la coscienza della sua vocazione europea, nei termini della sua Costituzione e sia perciò ancora capace di una preziosa opera di raccordo tra Paesi grandi e piccoli dell'Unione europea, tra Paesi fondatori e Paesi di nuova adesione, tra passato e futuro, tra interessi nazionali e interesse comune europeo». Grazie al nostro relatore; peccato che di tutto questo non vi sia traccia, all'indomani di Berlino e di Bruxelles, in nessuna dichiarazione dei Ministri del nostro Governo; peccato che il nostro Presidente del Consiglio abbia assistito alla demolizione di quell'edificio le cui basi anche noi italiani, tutti indifferentemente, avevamo contribuito ad erigere sulla scia dell'entusiasmo comune; peccato che il nostro Presidente del Consiglio sia rimasto impassibile, quasi indifferente. Come si dice in questi casi, davvero mai silenzio fu più assordante.

tra le deleghe contenute nella legge comunitaria e la delega complessiva che negli ordini del giorno presentati verrà data al Governo per la successiva fase

Nella nostra discussione è stato centrale il giudizio sulle conclusioni del Consiglio di Bruxelles, giudizio che ha avuto diversi accenti negli interventi del senatore Mantica, del senatore Filippi, del senatore Zanone, del senatore Santini

per quella che è stata una decostruzione di uno strumento giuridico che si era faticosamente costruito, cioè il Trattato costituzionale europeo. Ebbene io non smentirò certo questo senso di di delusione ma direi che ora dobbiamo guardare al futuro, non attardarci su quello che è stato il sia pure recente passato. Se si "ricostruisce" la decostruzione, magari con l'aiuto dello splendido *dossier* preparato dai nostri dai nostri Uffici, allora si capisce che i *leaders* europei a Bruxelles si sono concentrati concentrati su due obiettivi. Il primo obiettivo è stato di metodo: quello di abbandonare il peso di una terminologia di tipo costituzionale che avrebbe portato a pericolosi *referendum* nazionali. Non tutte le Costituzioni sono felici come la nostra che ha escluso, con l'articolo 75, la possibilità di un *referendum* su un trattato internazionale e l'ha escluso dal 1948, quindi in tempo non

viene ribadito attraverso la conferma di quella cooperazione strutturata in materia di difesa che costituisce un fulcro della nostra

inoltre, che il principio di libera concorrenza è uno strumento e non un obiettivo ha rappresentato una presa di posizione contro l'idea dell'Europa come cavallo di Troia della globalizzazione. No, l'Europa è un'altra cosa; l'Europa è fondata su un modello sociale che crede nella libera concorrenza, ma come strumento per un mercato aperto e non già come obiettivo.

e una costituzione materiale europea si è affermata anche se non si chiama così. Sul frontone del tempio di Apollo a Delfi c'era scritto: invocato o non invocato, il dio sarà presente. Ebbene, il "dio Costituzione" è presente, anche se non si chiama più con questo nome.

Signor Presidente, oggi come ieri, direi come sempre, come hanno intuito i nostri padri costituenti con l'articolo 11 della Costituzione, che ancora oggi è uno degli strumenti più agevoli in Europa per consentire il passaggio dall'ordinamento europeo a quello nazionale, l'interesse nazionale italiano coincide Ne abbiamo bisogno in ogni campo, sia che si parli di politiche spaziali - e dunque il progetto Galileo di Eufemi - sia che si parli di politiche sociali, come ha sottolineato il senatore Allocca. Ha ragione il senatore Girfatti quando dice che dobbiamo lottare e cercare

innanzitutto permettetemi di ringraziare tutti voi, senatori della maggioranza come dell'opposizione, per il lavoro svolto in Commissione e per il dibattito in quest'Aula, che credo abbia trovato, al di là di qualche elemento specifico, una grande concordia di fondo, almeno nelle linee da seguire, sia puntualmente per quanto riguarda la legge comunitaria vera e propria, sia sulla relazione, quindi sulle indicazioni di iniziativa politica. Consentitemi di cominciare da questa seconda parte, cioè dalla relazione, perché è a questa seconda parte più eminentemente di indirizzo politico che ha fatto riferimento la stragrande maggioranza degli interventi non solo stamattina, ma anche nella fase precedente del dibattito.

e certamente ha avuto anche elementi, come dire, di difficoltà. Il collega Zanone faceva riferimento - e molti lo avete fatto - ai simboli e all'importanza di quelli che sono stati cassati. È vero che non c'è neanche l'Inno di Mameli nella Costituzione italiana;

modo, l'intero vertice si è svolto con le bandiere con le stelle gialle che sventolavano ovunque - anche in quel caso sono sopravvissuti tutti - però poi

l'impronta intergovernativa rischi di avere una prevalenza eccessiva. Da questo punto di vista credo che

anche l'abbandono della concorrenza come obiettivo dell'Unione è avvenuto con una procedura piuttosto svelta. dobbiamo riconoscere al presidente Prodi e ad altri almeno l'intervento di stop per recuperare questa

farci prestare molta attenzione ai mesi che abbiamo di fronte. Per il resto, credo sia questa

Non mi unisco ai detrattori totali del processo di Barcellona, dico però che l'idea di Barcellona è del 1995 siamo nel 2007. È perciò probabile che anche l'idea nata a Barcellona necessiti di qualche aggiustamento: dato che si invecchia tutti, invecchiano anche le visioni, che non sono più all'altezza e adeguate al momento. Particolare rilievo, in questo senso, credo vada attribuita ad un'analisi serena - ripeto, serena - del *dossier* Turchia. Penso che il nostro Paese abbia un ruolo da giocare, proprio per eliminare quell'aspetto a mio avviso eccessivamente emozionale che ha accompagnato tutti i dibattiti sul processo di adesione della Turchia.

solamente una collocazione geografica e tanto meno solamente un'aderenza ad una singola religione. Da questo punto di vista, non ci nascondiamo le difficoltà che abbiamo di fronte, ma siamo anche convinti che, nel tribolato

e del clima. I parametri che sono stati accettati dai Capi di Stato e di Governo sono molto ambiziosi e credo che essere conseguenti significherà uno sforzo da parte di tutti, anche del nostro Paese,

uno sforzo diplomatico, affinché grandi Nazioni, grandi potenze che ancora non hanno accettato l'impostazione o l'impalcatura non solo del Trattato di Kyoto, ma addirittura dell'importanza di questo tema, si avvicinino con politiche convergenti. infatti che, se l'Europa resta da sola e non riesce a portarsi dietro Paesi come l'India, la Cina e gli Stati Uniti (per citarne solo alcuni), rischiamo di avere una politica certamente ambiziosa, ma forse non efficace agli obiettivi che ci siamo proposti, cioè quelli della riduzione delle emissioni, della riduzione dell'uso del petrolio, dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile. Lisbona il punto di riferimento delle politiche complessive per la crescita, come stabilite dall'Unione Europea, e credo che anche a tale proposito vadano il merito di aver iniziato a farli e di essere in linea rispetto ad alcuni dei capitoli previsti dall'Agenda di Lisbona, ma non ha mancato di sottolineare come rispetto ad altri capitoli gli sforzi non siano ancora sufficienti.

vero e proprio. In Commissione, il dibattito è stato molto approfondito. Abbiamo voluto questa volta che fossero presenti ai lavori di Commissione molti dei Ministri e dei Ministeri competenti per materia, in modo che anche la 14a Commissione avesse una possibilità di dibattito nel merito e non solamente procedurale.

ovviamente è legittimato ad avere le sue opinioni, ma vorrei fare chiarezza sui tempi e le procedure attraverso cui siamo arrivati a questo inserimento. hanno valutato positivamente la proposta di riduzione del termine di esercizio della delega proprio per evitare

Sono sempre tante, ma l'avvio della struttura di missione, il rapporto stretto con tutte le amministrazioni e, mi auguro, soprattutto il recepimento di questo cambio strutturale possono aiutare tutti noi a non rincorrere sempre, con grande affanno, i risultati che pure ci prefiggiamo. Senza entrare nel dettaglio (abbiamo avuto molte occasioni per farlo), il Governo ha accolto alcune obiezioni e resistenze di singoli colleghi e di singoli Gruppi. È vero che abbiamo accettato il ritiro di alcuni articoli relativi a materie che ancora non sono oggetto di infrazione; vorrei però che questa Camera fosse avvertita che è solamente un rinvio di tempi, quindi mi auguro che di qui alla prossima comunitaria si trovi il modo di risolvere nel merito i problemi posti e che abbiamo rinviato rispetto a questo strumento. I problemi esistono. Mi auguro che vorremo tutti insieme trovare il modo per risolverli. Altrimenti, è solamente un rinvio, in attesa di un'infrazione che rischia di essere sicura. nel dire che in allegato non ci sono solo tutte le direttive ma anche le infrazioni, e che è pronto ed in funzione il sito aperto al pubblico, in cui potrete potrete vedere l'andamento e le motivazioni delle infrazioni, e tenuto conto degli emendamenti che tratteremo più tardi e dell'ordine del giorno torno a ringraziare tutti per il lavoro svolto insieme. Mi auguro sia un passo avanti per un'accelerazione ed una maggiore credibilità del sistema del Paese in termini di compatibilità con gli ordinamenti comunitari.

la critica che rivolgiamo a questo provvedimento è inerente sostanzialmente - direi esclusivamente - all'articolo 31 e seguenti

Premetto immediatamente che non siamo contrari alle previsioni contenute in questo Capo, peraltro importantissime e che riguardano temi assai rilevanti, che contribuiscono a costruire quello spazio di libertà, giustizia e sicurezza che la riunione di Tampere nel 1999 aveva stabilito come cogente in materia di giustizia e affari interni. È noto che la nostra politica in Europa dal 2001 al 2006 si è differenziata dalle politiche precedenti (non so da quelle attuali, perché malgrado vi fosse un ordine del giorno che impegnava il Governo a riferire periodicamente alla Commissione giustizia sull'attività

si è differenziata soprattutto per il fatto che non abbiamo mai accettato quella pedissequa, e secondo me acritica, posizione per la quale tutto ciò che fa l'Europa è bene e quindi va e quindi va acriticamente approvato. Noi abbiamo cercato di distinguere il grano dal loglio, quindi di approvare i provvedimenti che a nostro avviso fossero condivisibili, diversamente da quelli che invece

vige ancora oggi finché non verrà approvata una Costituzione - il criterio dell'unanimità in Consiglio dei Ministri; quindi, era evidente che tali decisioni-quadro non avrebbero potuto mai essere approvate se non vi fosse stato anche l'assenso del Governo italiano,

e quindi, di fatto, in Commissione giustizia si è potuto semplicemente esprimere un parere, non esaminare queste norme, che sono fondamentali. Ricordo che parliamo di questioni non secondarie. Parliamo di introdurre un principio che nel nostro codice penale non c'è: quello della corruzione privata, che avrà conseguenze enormi da oggi in poi su tutto il sistema economico italiano. Stiamo parlando di questo, colleghi. Stiamo parlando dell'assunzione delle prove, della confisca di beni e quindi del fatto che in qualche modo cediamo un pezzettino di sovranità nazionale. temi che, ripeto, abbiamo condiviso, perché riteniamo riguardino questioni che giustamente vanno portate a livello europeo.

far rilevare che, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del reato di corruzione privata, viene scritta una delega di tre commi, patentemente ed evidentemente anticostituzionale.

sulla delega relativa all'introduzione del reato di corruzione privata; una delega su un tema assolutamente rilevante, attuata con tre commi.

riscritta in termini costituzionalmente corretti, esaminata e approvata, come è giusto e corretto che sia, dalle Commissioni competenti, cioè le Commissioni giustizia di Camera e Senato. Sono anche disponibile al ritiro questa proposta di non passaggio agli articoli nel caso che la mia posizione, soprattutto per quanto riguarda il reato di corruzione privata, venga presa in considerazione. Siamo assolutamente d'accordo sulla sostanza e sul contenuto, ma lo strumento

Signor Presidente, la questione è complessa. Tradizionalmente, come spiegava il collega Castelli, le decisioni quadro erano oggetto di un apposito provvedimento di legge dotato di tutti i crismi. Tradizionalmente, le decisioni quadro, assunte all'unanimità, ricadevano interamente nell'area cosiddetta intergovernativa e avevano la caratteristica di un accordo politico più che di un vero e proprio vincolo giuridico dello Stato italiano ad adottare un provvedimento. La situazione è cambiata

È possibile, cioè, passare dal sistema intergovernativo a quello comunitario (decisioni a maggioranza insieme con il Parlamento) attraverso un'opzione. Il Consiglio dei Ministri di giustizia e affari interni può decidere, all'unanimità, di rinunciare alla regola dell'unanimità e di passare alla regola comunitaria, ciò che peraltro, il Consiglio non ha finora mai fatto. Ciò è molto eloquente quanto alla serietà dell'impegno europeistico di molti Governi o alle difficoltà attraversate in questa ultima fase.

di comunitarizzare diverse aree, tra le quali, e prima di tutte, anche questa. Per quanto riguarda l'ordinamento interno italiano, la legge di riforma delle procedure di partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, che porta indegnamente il mio nome, si è azzardata a compiere un passo avanti. Noi abbiamo omogeneizzato la procedura di recepimento delle direttive e la procedura di recepimento delle decisioni comuni anche sulla base di un ottimismo, che si è poi rivelato parzialmente infondato e che adesso invece torna ad essere fondato, sulla prossima parificazione tra i due sistemi. Abbiamo cercato di realizzare un sistema normativo italiano che fosse all'altezza della futura costituzione europea, che adesso non sarà più una costituzione, ma che comunque ci sarà e che dovrebbe darci a breve la parificazione fra decisioni comuni

(anche le zucchine hanno a che fare con la libertà, ma non così direttamente). Non mi sento tuttavia di votare la proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Se invece il collega Castelli avesse avanzato un'altra proposta, se il collega Castelli avesse proposto di non passare alla discussione degli articoli perché il ministro Bonino non ha dato indicazioni chiare sulla linea politica del Governo, rifiutandosi di rispondere alle domande che le sono state rivolte in questa sede e ritenendo evidentemente più opportuno manifestare le sue intenzioni politiche ai giornali invece che all'Aula del Senato,

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi,

In quell'occasione ebbi già la possibilità di sollecitare l'attenzione dei colleghi su una questione giuridica, che però è anche una questione politica di grande momento e che rappresenta proprio la natura stessa della decisione quadro. Quest'ultima, secondo una dottrina piuttosto autorevole, sarebbe di per sé immediatamente applicativa, qualora i Paesi non addivenissero ad un'adesione nei tempi stabiliti.

il senatore Castelli ha ricordato che le decisioni quadro sono del 2003 e del 2005, quando l'attuale opposizione era al Governo. Allora l'Italia non presentò nessuna obiezione rispetto all'approvazione di queste decisioni quadro,

presentare delle riserve parlamentari, dicendo che la decisione quadro non avrebbe potuto essere adottata senza un'espressa approvazione da parte dei due rami del Parlamento. Collegavo tale questione al mandato di arresto europeo, perché in quella sede, oltre a svolgere la discussione, introducemmo una norma espressa nella legge che aderiva alla decisione quadro, stabilendo che ogni estensione della normativa sul mandato di arresto europeo potuto essere assunta dal Governo in sede europea solo previa riserva parlamentare, cioè con l'adesione esplicita preventiva del Parlamento italiano. Tale questione non è intervenuta in questa circostanza: la decisione quadro non ha nessuna riserva parlamentare ed è di per sé piena di quei criteri e principi direttivi che ne consentono

addirittura un secondo passaggio da parte del Governo, che dovrebbe rappresentante alle obiezioni delle Camere delle controdeduzioni, solo a seguito delle quali potrebbe essere formulata la legge delega.

Queste decisioni quadro non possono pertanto essere neppure modificate se andiamo a valutarne concretamente la sostanza. Aggiungo che, nonostante non sia intervenuta alcuna riserva parlamentare, la legge delega è lo strumento adeguato ed esclusivo. Credo che anche nel merito ci sia materia per discutere delle singole questioni. Mi riferisco a materie quali la corruzione, il sequestro e la confisca di beni, il riconoscimento reciproco delle sezioni amministrative; materie per le quali il nostro Paese certamente non avrà nessun problema

Gruppo di Alleanza Nazionale sostiene la proposta di non passaggio all'esame degli articoli presentata dal presidente Castelli (ovviamente con le subordinate che egli ha indicato), ritenendo veramente surreale la discussione in questo momento. Qualche giorno fa il Governo rischiava di cadere, per esplicita affermazione del Ministro della giustizia,

Su ciò la legge ordinaria veniva ritenuta un passaggio così importante da parte del Parlamento nazionale da incidere addirittura sulla stabilità del Governo. il Parlamento non avrebbe la possibilità di approfondire nelle sedi di merito - a cominciare dalla Commissione giustizia - questioni di tale peso, come una deroga a quella che è stata sempre la configurazione giuridica della corruzione da millenni (cioè la qualifica pubblicistica dell'agente) e le procedure di sequestro e confisca dei beni (che nel nostro ordinamento, peraltro, sono accompagnate e seguite da rimedi e impugnazioni che non hanno sempre eguali in altri ordinamenti europei ed esigono quindi un approfondimento in termini di armonizzazione).

proprio nel centro-sinistra ci si stracciava le vesti quando il Governo Berlusconi legittimamente poneva riserve e perplessità sull'estensione, al di là di ogni limite, del mandato di arresto europeo. Mi sembra veramente suggestivo che si capovolgano oggi i termini del discorso. Ad ogni modo, parliamo della questione per come essa si pone ora. Oggi ritengo fuori luogo che materie di diritto sostanziale e di diritto processuale di tale peso passino sotto il vaglio del Parlamento soltanto per un parere.

a dire la presenza in Aula a rappresentare il Governo, su un tema così rilevante, di un Ministro che ieri ha rassegnato le dimissioni o comunque rimesso il mandato (non si capisce bene che cosa sia successo) nelle mani del Capo del Governo.

alla loro situazione personale e per un senso di dignità della loro funzione. Qui, invece, le dimissioni sono collegate ad un fatto politico che in questo momento interessa l'intera Nazione, il Governo nel suo insieme ed il Parlamento: il futuro dei conti pubblici, sulla base dell'assetto che avrà il sistema pensionistico. Tutte queste ragioni, signor Presidente, credo facciano ritenere di buon senso l'appoggio alla proposta di

che in Commissione si è svolto un dibattito veramente notevole e contrastato su determinate posizioni del Gruppo

tra i reati presupposti dal suddetto decreto legislativo, ossia tra gli illeciti la cui commissione può determinare una responsabilità amministrativa da reato per le persone giuridiche, suscita perplessità, in quanto

l'impresa in via diretta ed autonoma, anche a prescindere dalla rilevanza penale dei comportamenti tenuti dalle persone fisiche, visto che la legislazione *antitrust* prevede un apparato sanzionatorio di estremo rigore. Le sanzioni pecuniarie per le imprese possono arrivare fino al 10 per cento del fatturato totale, oltre ad essere contemplate sanzioni di tipo interdittivo per le ipotesi di inottemperanza alle decisioni dell'autorità amministrativa competente, che è l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

e che quindi l'esistenza di un procedimento di fronte all'Autorità *antitrust* in nulla condiziona o limita la procedibilità di dette azioni e dei relativi procedimenti per l'affermazione della responsabilità penale delle persone fisiche. Da tutto ciò emerge - così come sottolineava anche il collega Castelli - che l'inserimento del reato di "corruzione nel settore privato" nell'ambito del sistema legislativo previsto dal citato decreto legislativo n. 231 non porterebbe ad una intensificazione della tutela dei soggetti lesi, ma certo determinerebbe il rischio di una sovrapposizione di piani e di tutele, con le conseguenti possibili ulteriori conseguenze: sanzionare due volte, ai sensi della legge *antitrust* ed ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, per il medesimo fatto o comportamento, a tutela del medesimo interesse giuridico (il mercato concorrenziale), le imprese italiane;

consiste nell'aggravio di costi per il sistema della giustizia nel suo complesso, ove si consideri che la responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231 del 2001 si accerta nell'ambito del processo penale.

Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterò a favore della proposta di non passaggio agli articoli, avanzata dal senatore Castelli. Naturalmente, se - come ha sollecitato anche il presentatore - il Governo fosse disponibile invece ad uno stralcio di questa parte, il problema non si porrebbe perché in realtà la questione - a parte i temi politici sollevati da chi mi ha preceduto - riguarda con precisione il Capo del disegno di legge che si riferisce all'attuazione di decisioni in materia penale.

anche altre parti del disegno di legge si sono giovate dell'occasione favorevole per veicolare, attraverso un Parlamento di difficile gestione, mi rendo conto, una serie di norme che forse non avrebbero

sul passaggio o meno agli articoli, il Ministro voglia dare un chiarimento, che, se fosse - come si diceva prima - nel senso della cancellazione o di uno stralcio di queste norme, forse consentirebbe una migliore veicolazione parlamentare della normativa,

si crea una normativa talmente aperta da ricordare molto il famoso abuso d'ufficio che si poneva per i pubblici dipendenti, cioè un meccanismo per poter sanzionare qualunque cittadino a prescindere

dove si fa riferimento alla previsione di adeguate sanzioni pecuniarie interdittive, addirittura in norma penale, laddove esiste un principio preciso di riserva di legge, si lascia ad un potere di secondo livello decidere anche la sanzione, violando apertamente i diritti di libertà dei cittadini, cosa che mi sembra non si possa fare se non appunto mediante un meccanismo di riserva di legge. E qui passiamo alla seconda parte dell'argomentazione: dell'argomentazione: l'articolo 30 definisce una procedura che si basa su un meccanismo di parere parlamentare al Governo. Qui si realizza la vera e propria violazione del principio di riserva di legge, perché un conto è decidere da parte del Parlamento le norme in materia penale,

difforme dal contenuto del testo governativo; ciò nondimeno, però, il Governo va avanti per la propria strada, creando un conflitto con il Parlamento (quindi, venendo in conflitto con l'organo legislativo) e, ciò nonostante, decidendo in materia penale,

vita comune. In secondo luogo, comunque, ogni norma che sanziona le libertà dei cittadini ha una sorta di sacralità giuridica che non può essere delegata ad un'occasione o ad un'istanza di secondo livello rispetto al potere legislativo. D'altronde, signor

Se non gli resta almeno l'esame delle norme fondamentali - come lo sono quelle relative alla convivenza civile, cioè, in primo luogo, il diritto penale - penso che il Parlamento abbia poca ragione di continuare a sopravvivere.

Presidente, sarei favorevole al passaggio agli articoli. Il Titolo III corrisponde - come hanno ricordato i senatori Buttiglione e Sinisi - ad un preciso obbligo della legge comunitaria. La materia è stata oggetto di un'ampia trattazione in sede di Commissione giustizia, con un parere che figura agli atti all'inizio del nostro fascicolo. La corruzione privata è certo una configurazione nuova nel nostro sistema penale, ma è esattamente prevista dalla Direttiva, la quale prevede anche le sanzioni per le persone giuridiche. Credo vi sia anche un'urgenza di provvedere a questo problema, perché nelle recente decisioni di Bruxelles si è posto l'accento sulla necessità di accelerare la comunitarizzazione delle norme penali. Concluderei con una nota non tecnica: temo che, se passasse il messaggio che il Senato ha accantonato la discussione sulla corruzione privata, privata, ciò avrebbe all'esterno della nostra Aula un significato devastante, sia per la nostra maggioranza sia - credo - per tutto il Senato.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: in ordine all'articolo 18, il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 18.200; in ordine all'articolo 28, il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al comma 2, primo periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)"*, sia eliminata la lettera nonché a condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, che siano inserite infine le parole "Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". In ordine agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.9, 5.0.100 e 8.103. In ordine alla proposta 1.30, il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che le parole: "all'articolo 2" siano sostituite dalle parole: "all'articolo 1". Sulla proposta 27.100 il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 27, comma 2, le parole "della delega di cui al comma 1" siano sostituite dalle parole "delle deleghe di cui al presente articolo". Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.0.100 e 5.0.60. Esprime parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.0.9 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che nel capoverso 4-*bis*, nell'ultimo periodo, prima delle parole: "il numero delle unità di personale viene stabilito" siano inserite le seguenti: "Nell'ambito del suindicato contingente," nonché a che siano soppressi i capoversi 4-*ter* e la lettera «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 27.100 (testo 3) relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

che hanno già previsto in sede di bilancio 2007 interventi ambientali atti a superare le procedure di infrazione comunitaria, di stanziare risorse disponibili in cassa ma non erogabili, secondo quanto previsto dalla sperimentazione sul Patto di stabilità per le Regioni definito nell'ultima legge finanziaria. Nella sostanza, la finanziaria limita al 25 per cento l'erogazione di risorse regionali, pur disponibili, a enti terzi: nel caso a cui si riferisce l'emendamento, alle Province. Segnalo al Governo come l'emendamento corrisponda in maniera puntuale allo spirito del disegno di legge; infatti, nella relazione tecnica si legge che il si legge che il mancato recepimento delle norme del disegno di legge (penso questo valga anche per le Regioni) provocherebbe «un reale rischio di esporre l'erario al maggiore danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di giustizia, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari». L'emendamento 2.0.100 va proprio nella direzione di permettere alle Regioni di non essere oggetto di sanzioni.

Tale relazione recita infatti: «Tale norma agisce come clausola di salvaguardia del sistema». Mi risulta infine che il fondo di rotazione a cui si riferisce appunto l'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, sia capiente in quanto già finanziato. Chiedo quindi al Governo di considerare attentamente questo emendamento.

Presidente, nel momento in cui il senatore Albonetti ha dichiarato di volere ritirare l'emendamento, ho fatto cenno alla Presidenza che desideravo intervenire. Lei mi ha dato la parola quando ha ritenuto di farlo, ma io ho appreso della volontà di ritirare l'emendamento solo pochi secondi fa.

al Governo nazionale, ma soprattutto in capo agli enti locali e alla Regione. In effetti, questo emendamento è incompleto per la non contabilizzazione nel Patto di stabilità

elaborato) estendere l'esenzione dal computo nel Patto di stabilità anche agli enti locali, che sono forse ancor più gravati delle Regioni per interventi straordinari in materia ambientale, e quindi possono ancor più risentire

si fa sempre più carico alle autonomie locali - e quindi anche alle Regioni - di interventi in materia ambientale, si deve intervenire sul Patto di stabilità riguardo a questo tipo di spese. Non si può pensare

Signor Presidente, vorrei farle presente un episodio singolare che è avvenuto in Commissione.

Dal resoconto sommario di quella seduta della Commissione, risulterebbe che questi due emendamenti del Governo siano stati respinti dalla Commissione. Ciò non è assolutamente vero, forse c'è stato un refuso. Allora era presente non il ministro Bonino ma il sottosegretario Li Gotti, il quale, appunto leggendo il parere della Commissione bilancio, ha ritenuto opportuno ritirare questi emendamenti. lei mi insegna, signor Presidente, che quando un emendamento viene ritirato in Commissione, in corso di esame della legge comunitaria dell'anno, non lo si può ripresentare in Aula, neanche con un altro tipo di testo. testo. Vorrei sottoporre alla sua attenzione questo increscioso fatto che si è verificato, anche perché capisco che abbia avuto il parere favorevole, pur con le modifiche proposte, ma mi sembra assolutamente - se mi permette il termine - non corretto aver ripresentato un emendamento quale il 5.0.100, che è assolutamente una marchetta plateale. Lo stesso - anzi vorrei la conferma dal collega Angius che mi era vicino in Commissione

A volte mi vengono in mente idee che non condivido che, però, riesco a combattere. Ma non riesco a combattere contro la pretesa autonomia del mio sistema elettronico. Ovviamente la mia vuole essere una richiesta di verifica di questa incongruenza.